specializzato nella produzione di elettrodomestici. La situazione dell'azienda era precaria già dal 2012 e lo stabilimento, già in procedura concorsuale, aveva ridotto la propria attività, proprio per problemi di liquidità,

Tutto ciò per una grave e continua mancanza di liquidità che aveva portato la situazione a precipitare, anche in seguito a un successivo e continuo diniego da parte degli istituti di credito

luce fra l'altro di un programma e di una consolidata capacità di produrre e di dare lavoro, mantenere vivo un tessuto economico importante come quello del bellunese.

ciò sia fondamentale per dare risposta a un territorio. Il commissario straordinario ne ha dato prova subito, aggregando le realtà del territorio: lavoratori, rappresentanti sindacali,

dai senatori Santini e Piccoli colgono un tema di grande rilievo e di importanza cruciale per l'area del bellunese. La ACC Compressors, come ricordano gli interpellanti, è un'azienda nata da uno *spin off* di Electrolux. Attualmente le quote della società sono detenute da fondi d'investimento che hanno deciso di non procedere alla necessaria ricapitalizzazione, e negli atti di sindacato si fa riferimento anche a questo che è un punto cardine della vicenda. L'intervento finanziario verso 1'ACC è assolutamente necessario per far fronte al rilancio della società a seguito delle vicende riportate dagli onorevoli interroganti, determinato tra l'altro il distacco della unità austriaca di ACC. Tale separazione ha ulteriormente indebolito la posizione finanziaria dello stabilimento di Mel. Per far fronte a tale indisponibilità da parte dei fondi proprietari a procedere alla ricapitalizzazione l'attuale gruppo dirigente si è attivato per individuare una soluzione societaria che prevedesse la partecipazione di una significativa parte dei creditori e l'impegno degli stessi a trasformare una parte del loro credito in *equity* e a finanziare la società con nuova liquidità.

Nella giornata del 3 giugno il Ministero è stato informato che una parte dei nuovi soci non aveva presentato la formale adesione al progetto, con ciò determinando la rinuncia anche degli altri sottoscrittori e facendo decadere questa ipotesi che pure poteva avere un rilievo importante per consentire una ripresa della ACC. A questo punto, alla fine del mese di giugno la ACC ha adito il tribunale di Pordenone affinché dichiarasse l'insolvenza della medesima società ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 270 del 1999, recante la disciplina della amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi. Accertata l'esistenza dei requisiti di legge, il tribunale ha dichiarato l'insolvenza della ACC in data 28 giugno nominando commissario giudiziale, su designazione del Ministro dello sviluppo economico, il dottor Maurizio Castro. Sulla base della relazione predisposta da quest'ultimo, con decreto in data 27 agosto 2013, il tribunale di Pordenone ha dichiarato l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria della ACC e, da ultimo, con decreto in data 4 settembre 2013,

Naturalmente l'obiettivo che il commissario è chiamato a perseguire è prima di tutto quello di mettere in sicurezza la prosecuzione dell'attività e dei rapporti di lavoro dell'azienda e cercare poi soluzioni che possano consentire di avere un futuro produttivo e occupazionale adeguato per la ACC. A questo scopo il commissario straordinario dovrà predisporre entro 60 giorni dall'apertura della procedura, il programma di prosecuzione delle attività dell'impresa, con le relative previsioni economico-finanziarie, le connesse modalità di copertura del fabbisogno e le concrete ipotesi di sbocco futuro della procedura.

interpellanti quali sono le prospettive che si determineranno alla luce del piano stesso. Per quanto concerne la situazione occupazionale, il Ministero del lavoro ha il Ministero del lavoro ha seguito la vicenda e il 10 settembre 2012 la società ACC e le organizzazioni sindacali di categoria hanno sottoscritto un verbale di accordo che prevede, anche al fine di ridurre l'impatto occupazionale delle misure di ristrutturazione, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria «per ristrutturazione per complessità dei processi produttivi» a decorrere dal 13 ottobre 2012, per la durata di dodici mesi.

che ne prevede l'utilizzo per tutta la durata dell'attività del commissario (e quindi in base al programma che poi il commissario stesso presenterà). Continueremo quindi a seguire con grande attenzione la vicenda della ACC che - ripeto - è molto importante sicuramente per il territorio bellunese, ma anche per l'intero settore dell'elettrodomestico nel nostro Paese e, alla luce del

credo che sia davvero molto importante riuscire a supportare l'azione del commissario, che sembra già essere abbastanza efficace sul piano del recupero dei volumi produttivi.

Il problema, come ha sottolineato la collega Bellot, riguarda il fatto che naturalmente questo impatta con le esigenze finanziarie e di liquidità, in particolare di risorse per sostenere questo volume di produzione, perché, data la situazione dell'azienda, naturalmente i fornitori

la possibilità di costruire l'ingresso di possibili nuovi soci, di individuare *partner* sia commerciali, sia produttivi, in un mercato che è difficile, ma in cui, per la sua storia e per la sua qualità, questa azienda ha una posizione di *leadership*, certamente appannata negli ultimi anni, ma ancora ricostruibile, se riuscisse a dispiegare in pieno le sue facoltà. Questo naturalmente avrebbe effetti

in tempo debito, ma ovviamente noi vorremmo che fossero usati il meno possibile, cioè che il più rapidamente possibile si tornasse ad avere l'intera occupazione all'interno dell'azienda. Ma, perché questo succeda, servirebbero questi due interventi specifici, oltre al quadro generale strategico qui rappresentato, IVA e una linea di credito robusta, che permettessero di sostenere lo sforzo produttivo che in questi mesi si sta rendendo rendendo possibile e che sembrerebbe anche essere di ottime dimensioni. Mi fermo qui. Naturalmente ci sono tutte le osservazioni che la collega ha fatto e che io ripropongo sulla sulla velenosità dell'utilizzo finanziario delle presenze dentro le aziende. Quest'azienda paga l'uso speculativo di fondi finanziari che non hanno badato minimamente alla produzione, ma hanno badato solo a spremere le possibilità

Signora Presidente, ringrazio il Sottosegretario, che così puntualmente e in modo sintetico ha riassunto una storia che è davvero complicata. Riporto il punto della mia interrogazione: produzione strategica per il bellunese, ma produzione strategica anche per l'intero Paese. in Veneto possediamo, credo a vantaggio di tutta l'Italia, dell'intera filiera (dall'università allo sviluppo, alla ricerca) che riguarda la produzione di di compressori, il cuore strategico della tecnologia del freddo. Chiedevo di sapere quali fossero i possibili interventi a brevissimo, a medio e a lungo termine. Mi soffermo brevissimamente sulla risposta, formulando anche ulteriori richieste al Governo. La prima è di carattere generale. Mi pare ‑ come è stato detto poco fa ‑ che sia piuttosto evidente come sia necessario promuovere azioni di seria vigilanza in merito alle modalità con le quali i fondi d'investimento di profilo esclusivamente finanziario operano, dimenticando l'orientamento e la vocazione industriale, dal contenuto anche rilevante (com'è il caso in esame) delle nostre aziende, depauperandole e svuotandole. Quindi, credo che il pubblico debba porsi il problema dei modi con cui controllare queste attività. Il caso della ACC di Mel è quello di un'azienda che, in dieci anni, è stata letteralmente svuotata di capacità e di autonomia finanziaria. Quindi, vi propongo di immaginare qualcosa - uno strumento legislativo - che permetta, nei limiti della libera intrapresa di ciascuno, di controllare queste modalità. Anche perché, rimanendo nell'ambito della provincia di Belluno, spostandosi solo di qualche chilometro, in questi giorni sta divenendo evidente il caso di Ideal Standard, produttore di

rimesso in gioco, per ragioni che mi sfuggono, ma che certamente attengono agli interessi del fondo di investimento che lo possiede. Il tema è quindi particolarmente importante. Trascuriamo il fatto locale e allarghiamo il *focus*: è un tema di interesse per l'intero Paese.

produttive: gli istituti di credito, infatti, non concedono qualche milione di euro di liquidità a brevissimo. Questo potrebbe davvero compromettere il rilancio dell'attività strategica per l'intero Paese. Dico anche, come comunicazione, che il territorio non è stato a guardare. Ad, esempio nella fornitura del gas, grazie alla presenza dei Comuni in un grosso *player* nazionale, è stato possibile ottenere delle condizioni a prescindere dalle garanzie. Quindi questo è sempre nel novero della possibilità finanziaria dell'azienda. Mi associo alla richiesta di sbloccare questo credito IVA, perché è davvero importante. Non è stato detto, e lo aggiungo come dato, che lo stipendio di

relazione al quale gli interpellanti hanno manifestato la necessità di dare respiro e di permettere, quindi,

Signora Presidente, colleghi, interroganti, prima di affrontare nel merito la questione posta con l'atto di sindacato ispettivo, soffermarmi brevemente sull'importante e indiscusso ruolo che l'Arma dei carabinieri svolge nell'ambito dell'ampia missione affidata alle Forze armate per la difesa del Paese e la salvaguardia delle libere istituzioni. Come sapete, l'Arma non solo concorre alla difesa integrata del territorio nazionale, ma partecipa anche alle operazioni per il mantenimento e il ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale, contribuisce alle attività volte alla ricostruzione e al ripristino dei corpi di polizia locali nei teatri operativi, garantisce i servizi di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero ed esercita le funzioni di polizia militare, in via esclusiva per tutte le Forze armate. Fatta questa premessa, per quanto concerne l'opportunità di accorpare le stazioni dei Carabinieri di Sant'Agata de' Goti, Dugenta e Telese Terme - come auspicato dal senatore interrogante - sottolineo che tali stazioni, competenti sugli omonimi Comuni e, rispettivamente, su quelli di Durazzano, Limatola e Castelvenere, non sono incluse in alcuno dei progetti, dei progetti, recentemente avviati dall'Arma dei carabinieri, di razionalizzazione del dispositivo territoriale e non risultano, allo stato, interessate da altre proposte ordinative; ciò in considerazione della riconosciuta e indubbia funzionalità dell'attuale assetto istituzionale operante nell'area geografica interessata. Prima di concludere, vorrei quindi porre in risalto - e rassicurare il senatore - come l'Arma dei carabinieri abbia sempre posto notevole e costante attenzione nel perseguimento di un dispositivo territoriale efficiente e adeguato adeguato per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, tra cui quello della tutela della sicurezza dei cittadini e del territorio.

poiché il ruolo dei nostri Carabinieri va ricordato, e certamente l'Arma dei carabinieri ha sempre posto notevole e costante attenzione al perseguimento al perseguimento di un dispositivo territoriale efficiente ed adeguato (i nostri ragazzi lavorano per noi e per la Patria). Tuttavia, noto che tali premesse hanno occupato metà dell'intervento. La La sostanza propria della risposta, quindi, non solo è breve rispetto all'ampiezza formale dedicata, ma anche proprio nella sua stessa sostanza.

noi siamo semplici portavoce: non siamo venuti qua per fare quello che pensiamo noi o ciò che pensa eventualmente il partito, ovvero cinque persone che si chiudono in una stanza. No, noi siamo i portavoce dei cittadini, e i cittadini di quella zona chiedono, ancora una volta, al Ministro - e a gran voce che vengano presi dei provvedimenti e l'accorpamento delle stazioni dei Carabinieri di Dugenta (Benevento), Telese Terme (Benevento) e Sant'Agata dè Goti, in modo da istituire una tenenza dei Carabinieri a Sant'Agata de' Goti, che avrebbe proprio il compito di svolgere le funzioni di polizia nei Comuni di Dugenta, Durazzano, Sant'Agata de' Goti, Limatola, ad esclusione della stazione di Telese Terme, in quanto è già presente un commissariato di polizia. Questo garantirebbe una maggiore sicurezza dei cittadini. Se invece il Ministro non ritiene sembra, avviare tale processo di razionalizzazione del dispositivo territoriale, perché attualmente non previsto, a questo punto i cittadini chiedono l'eliminazione delle scorte - se ci sono ancora - degli ex Presidenti di Camera e Senato e una riduzione drastica delle scorte per i Ministri, i parlamentari e i Presidenti di Camera e Senato, per impegnare così la somma risparmiata nell'incremento della sicurezza dei semplici cittadini, che pagano tasse molto alte e hanno il diritto di godersi in

si sono introdotti in uno stabile con due abitazioni occupate da due sorelle e, dietro minaccia, hanno costretto le vittime a farsi consegnare oro, soldi, due televisioni e altrettanti *personal

a via Sant'Antonio Abate, a bordo di una monovolume Renault Scénic, hanno rubato 20 bombole di GPL dal deposito di una rivendita per prodotti agricoli, ubicata di fronte all'istituto di istruzione superiore «Sant'Alfonso Maria de' Liguori». Il commerciante santagatese, abitante nei pressi del magazzino, svegliato dai rumori, ha urlato dal balcone mettendo in fuga i due balordi. Qualche

I cittadini chiedono normalità, null'altro.

in via preliminare faccio notare che, a carattere generale, la questione relativa all'intervento in chiave riduttiva delle unità da reclutare nell'ambito del concorso richiamato dal senatore Cardiello è stata già affrontata di recente in risposta ad un atto dell'onorevole Rosato. Pertanto, come già rappresentato nell'ambito della predetta risposta, non posso che confermare che tale questione deve porsi in relazione alla stringente necessità di pervenire a risparmi per effetto della cosiddetta *spending review*,

Conseguentemente, è stato inevitabile per questa amministrazione intervenire drasticamente, operando un indispensabile ridimensionamento ridimensionamento delle spese relative al settore del personale della Difesa, con conseguenti ripercussioni anche sull'entità complessiva dei reclutamenti previsti nel 2012, per l'esercito, la marina e l'aeronautica. Tale intervento in chiave riduttiva evidentemente ha interessato, in varia misura, anche il reclutamento del personale dei diversi ruoli delle Forze armate, tra cui anche i volontari in ferma prefissata quadriennale, i cosiddetti VFP 4. Nel merito, si ribadisce che con tale intervento - peraltro rientrante nella facoltà dell'amministrazione, così come previsto nel bando concorsuale - si è inteso, tra l'altro, guardare anche in prospettiva, nel senso di salvaguardare, il più possibile, il personale coinvolto, immettendo in ferma quadriennale un numero di unità tali da consentire alle stesse adeguate possibilità di transito nei ruoli del servizio permanente. Ciò premesso, venendo alla presunta mancata immissione dei vincitori del concorso indetto per il 2012, rassicuro il senatore Cardiello che, secondo le indicazioni del competente Stato maggiore dell'esercito, tutti i 2.075 VFP 4 vincitori sono stati regolarmente incorporati nelle Forze armate. Ciò è avvenuto attraverso due distinti momenti di immissione, rispettivamente in data 21 agosto 2012

comportato anche la ridefinizione delle tempistiche delle successive fasi di selezione e incorporazione dei candidati.

ci sono migliaia di ragazzi che hanno promosso un ricorso al tribunale amministrativo del Lazio per poter ottenere un'ordinanza o, eventualmente, una sentenza affinché il Ministero della difesa ottemperi all'assunzione di questi ragazzi.

da zone tristemente note per l'alto tasso di criminalità organizzata, e questi ragazzi che nutrono una speranza per il futuro e partecipano ad un concorso secondo me non possono essere trattati in questo modo. Le dico io le cifre del concorso quanti e quali sono stati assunti nelle Forze dell'ordine, perché a volte si finisce nel ridicolo. Il Ministero della difesa nell'ottobre del 2011

più facile far scorrere la graduatoria e chiamare in servizio questi ragazzi? Quindi, signor Sottosegretario (so che in questo momento ci stanno guardando migliaia di ragazzi, perché, come lei sa, sul *web* ci si passa la voce), mi auguro che il Ministero della difesa possa assumere un impegno nei confronti dei ragazzi che sono stati dichiarati idonei e attendono una risposta nell'immediato.